ieri è scomparso Luigi Preti e vorrei ricordarlo all'Assemblea nella sua attività. il senatore Vizzini ha chiesto di parlare sull'ordine dei lavori anticipando l'argomento. consentire al senatore Vizzini il suo intervento, anche se non attinente ai provvedimenti all'ordine del giorno, perché riconducibile a quella casistica di eventi straordinari che, unanimemente, abbiamo

politico di grande qualità, uomo di cultura, autore di numerose pubblicazioni. Luigi Preti da giovane svolse attività antifascista e fu costretto a ritornare in Svizzera, rientrando in Italia dopo l'8 settembre del 1943. *(Brusìo).*

e più volte Ministro, Presidente del Gruppo socialdemocratico alla Camera dei deputati, Vice presidente della Camera, Presidente del Partito Socialista Democratico Italiano, anche nel tempo in cui io fui segretario politico di tale partito ed ebbi l'onore di lavorare al suo fianco. Luigi Preti è stato un riformista moderato, che nella sua vita ha combattuto il fascismo ed il comunismo, lavorando alla costruzione di un'area socialista democratica riformista in tutti i modi in cui fu possibile nella stagione della sua attività politica. Lo ricordo anche nel Partito Socialista Unificato, alla fine degli anni '60, come *leader* e componente della corrente autonomista di quel partito. La caratteristica che ricordo di lui nella sua azione di uomo di Governo è quella di un uomo che ha sempre avuto il senso dello Stato. volte Ministro delle finanze ed avviò una riforma tributaria, sulla cui impalcatura ancora si regge il nostro Stato, ma fu anche Ministro dei trasporti e della marina mercantile e Ministro del bilancio. alla crescita della nostra Repubblica e dello Stato democratico e, dietro la sua figura fisica di uomo minuto, vi sono sempre state grandi idee, forza per la vita della democrazia italiana. Lo ricordo come uomo che si è sempre battuto per la libertà e la giustizia sociale come fondamenti e cardini ineludibili di una grande democrazia occidentale, quale quale è stata l'Italia nel periodo della sua attività politica. Credo che tutte le compagne ed i compagni socialisti democratici d'Italia lo ricorderanno sempre nei loro cuori, con il dolore di averlo perso. Vorrei portare alla famiglia il sentimento di un cordoglio vero per aver perduto un grande italiano.

che in questo Paese, quando sono state fatte le battaglie per la libertà, per l'emancipazione dei lavoratori, degli operai e degli ultimi, ha dato un grande contributo. Quindi, poche parole per

Luigi Preti. Ne ricordiamo la funzione importante che ha avuto all'Assemblea Costituente ed il ruolo importante che da socialdemocratico ha svolto per una spinta critica e riformista a sinistra, contribuendo anche a contribuendo anche a far sì che questo Paese fosse, anche dal punto di vista sociale, più moderno e più adeguato ai bisogni dei cittadini. Signor Presidente, anche il Gruppo della Lega Nord si associa al cordoglio ed al ricordo di Luigi Preti. Socialdemocratico, lo si ricorda per alcuni

da radicalismi e massimalismi. Quindi, anche da parte nostra ci associamo al ricordo e al cordoglio per questa persona che ha lavorato tanto per il nostro Paese.

Vizzini e ritiene che il Paese perda una figura non solo di grande spessore politico e culturale, ma anche espressione di una cultura, quella riformista, che ha dato un grande contributo allo sviluppo, all'evoluzione della democrazia del nostro Paese e alla vita delle istituzioni repubblicane. Il Governo quindi si associa al cordoglio alla famiglia.

seppur brevemente, di anticipare quello che sarebbe stato l'oggetto del suo intervento, in particolar modo la richiesta - che lei avrebbe fatto - di un cessate il fuoco sulla vicenda di Gaza. Quindi, il suo intervento sull'ordine dei lavori non non le è stato consentito compiutamente, ma nella prima fase lei ha avuto modo, attraverso il consenso della Presidenza, di anticipare quella che poi non è stata altro che una sintesi del successivo intervento

costituisce una tappa fondamentale del suo percorso verso la valorizzazione delle autonomie territoriali e la responsabilizzazione delle relative classi dirigenti, in una prospettiva che assicuri comunque un adeguato sostegno alle aree territoriali in ritardo di sviluppo e che, proprio per tale motivo, necessitano di un intervento pubblico adeguato e qualitativamente superiore alle altre aree, indipendentemente dalla capacità di farvi fronte con la propria capacità fiscale. Un dato fattuale che appare in sé significativo, alla base dell'intervento normativo in commento, è quello che mette in evidenza come, nella generalità dell'opinione pubblica, nonostante la complessità dell'argomento e la retorica che spesso ne ha inquinato il dibattito, si stia acquisendo la consapevolezza che il federalismo fiscale costituisce anzitutto una riforma indispensabile per combattere l'inefficienza delle amministrazioni pubbliche e aggiornare, così, alcuni elementi del «patto fiscale» tra istituzioni e cittadini. Un sistema di finanza derivata, come dimostra la teoria e come si è acclarato sulla base della stessa evidenza dei fatti, che operi con ripiani a piè di lista in favore delle amministrazioni inefficienti, ovvero con criteri basati prevalentemente sulla spesa storica, finisce infatti spesso per premiare chi più ha creato deficit, favorendo comportamenti che creano disavanzi destinati prima o poi ad essere coperti dalle imposte a carico di tutti gli italiani. In termini più semplici, un sistema di finanza derivata finisce per consacrare il principio per cui chi ha più speso in passato può continuare a farlo, mentre chi ha speso meno - perché è stato più efficiente - deve continuare a spendere meno. In proposito, la sfida del federalismo starebbe pertanto nel contributo che esso dà alla partecipazione democratica ed al controllo dei cittadini sulla cosa pubblica, nonché nel processo di concorrenza emulativa tra comunità e governi locali in un contesto di responsabilità. Passando all'esame del testo, va tenuto preliminarmente conto del fatto che alcuni aspetti della proposta scontano il mancato adeguamento dell'assetto costituzionale. È chiaro il Senato federale delle Regioni sarebbe stata forse una sede ancor più idonea per esaminare tali aspetti. Nel suo complesso, l'intera architettura della delega appare comunque conforme al modello costituzionale vigente, seppure le ricadute concrete della sua implementazione saranno apprezzabili solo con i decreti di attuazione. Questi erano e rimangono i capisaldi che ispiravano il testo inizialmente proposto dal Governo. Ma l'esame da parte delle Commissioni riunite ha modificato in profondità quel testo accogliendo molte sollecitazioni, alcune presentate anche dalle opposizioni. Per questo motivo, in questa prima parte illustro le linee portanti del provvedimento così come approvato dalle Commissioni riunite, rinviando alla successiva parte la disamina di dettaglio di tutte le modificazioni apportate nel corso dell'esame da parte delle Commissioni riunite. Venendo in particolare all'esame degli aspetti concernenti la coerenza del disegno di legge con l'impianto costituzionale del Governo della finanza pubblica, va dato preliminarmente conto dei numerosi correttivi apportati già in sede di affermazione dei principi generali. Tra questi basti citarne, tra i tanti, almeno due. Un primo elemento di sicuro rafforzamento della «civiltà giuridica» tributaria è rappresentato dall'introduzione, all'articolo 2, dei principi generali della semplificazione del sistema tributario, della riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, della trasparenza del prelievo, dell'efficienza nell'amministrazione dei tributi, del coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, del rispetto dei principi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente. Un secondo punto qualificante nell'ambito dei principi generali è l'affermazione del principio della certezza delle risorse e della stabilità tendenziale del quadro di finanziamento, in misura corrispondente alle funzioni attribuite. Venendo alla disciplina più specifica della nuova configurazione dei rapporti finanziari tra i livelli di governo, va segnalata la previsione della armonizzazione di tutti i bilanci pubblici. Di altrettanta rilevanza è l'introduzione del patto di convergenza nel testo approvato dalle Commissioni, congegnato a regime e ben precisato nei suoi termini di funzionamento. Sul piano delle fonti di finanziamento, il disegno di legge definisce i lineamenti di un quadro diretto a permettere l'esercizio concreto dell'autonomia tributaria da parte dei governi decentrati, prevedendo, in particolare, che le Regioni possano istituire tributi propri ma solo per i presupposti non già assoggettati a imposizione erariale. Il testo assicura altresì un adeguato livello di flessibilità fiscale nello sviluppo del disegno complessivo di federalismo, attraverso la previsione

dal modello emerge la rilevanza della scelta di distinguere le spese che investono i diritti fondamentali di cittadini separatamente rispetto a quelle che, per il loro minore significato equitativo, vengono affidate in misura maggiore al finanziamento con gli strumenti propri dell'autonomia tributaria e, perciò, nel limite della capacità fiscale degli enti decentrati, pur con il sussidio anche in questo caso del fondo perequativo. auspicabile che tali criteri siano resi il più possibile chiari e trasparenti in sede di attuazione della delega. delega. Il tema dell'individuazione e della delimitazione dell'ambito delle funzioni riconducibili ai diritti civili e sociali (spese fondamentali) è pertanto ovviamente cruciale. Nel corso dell'esame delle Commissioni riunite, in proposito, è stato chiarito che l'indicazione delle tre funzioni essenziali, dal Governo individuate in sanità, assistenza e istruzione, è invece da intendersi riferita alle spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, lettera *m)*, della Costituzione. Aspetto distinto, invece, è quello della definizione, anche questa cruciale, dell'ambito definitorio di tali funzioni essenziali, aspetto che sarà definito dalla normazione delegata. Un capitolo a sé stante, di evidente, rilevantissimo valore, è quello della corretta determinazione dei costi standard delle spese corrispondenti alle funzioni fondamentali. Anche questo punto è stato oggetto di approfondimento e il testo approvato ha chiarito che il costo standard è quello che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto a cui comparare e valutare l'azione pubblica. Ai fini della puntuale definizione dei parametri per la stima dei predetti costi standard, la norma richiamata specifica infatti che l'erogazione delle prestazioni essenziali deve avvenire in condizioni che assicurino comunque la «efficienza ed appropriatezza» su tutto il territorio nazionale. Anche in questo caso, si tratta di norme di principio condivisibili, tenuto conto in particolare delle esperienze in tema di spesa sanitaria. Si segnala inoltre che il testo stabilisce espressamente che la definizione degli strumenti della fiscalità derivata, per le Regioni, dovrà essere fissata ad un livello minimo, tale comunque da assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle delle prestazioni in «una sola Regione» e non in «almeno» una Regione, come nel testo del Governo, fermo restando l'accesso alla perequazione per tutte le altre, con ciò significando che, per le Regioni che non risulteranno comunque autosufficienti, si provvederà si provvederà con un trasferimento dal fondo perequativo, finanziato attraverso la compartecipazione all'IVA, che consentirà di finanziare integralmente i loro fabbisogni. È chiaro che, con ogni probabilità, l'unica Regione in grado di soddisfare queste istanze di chiarezza risulterà quella che ha la maggiore capacità fiscale, conseguendone che la compartecipazione verrà fissata ad un livello percentuale relativamente basso, che, per i fabbisogni delle altre Regioni, vorrà dire l'accesso al sistema di perequazione. Va da sé che l'individuazione di questo paniere di aliquote, se soddisferà la corrispondenza tra tributi, capacità fiscale e fabbisogni in una Regione, porrà le altre Regioni in una posizione più favorita, ovvero nella necessità di dover ricorrere al fondo di perequazione. Pertanto, tanto più bassa sarà la percentuale media di compartecipazione ai tributi adottata, in relazione all'esigenza di consentire l'autofinanziamento dei servizi essenziali da parte di almeno una Regione, tanto maggiore sarà l'eventualità di attivare la perequazione per le altre. Tutto dipenderebbe, in tale schema, dalla Regione assunta a parametro e dalla sua «capacità fiscale». In proposito, è stato chiarito anche il punto relativo alla collocazione del finanziamento della spesa per il trasporto pubblico locale, per il quale si è previsto che l'attribuzione delle quote del fondo perequativo sia subordinata al rispetto di un livello di «servizio minimo». Per le altre competenze, invece, il concetto di fabbisogno standard non viene adottato in quanto, per queste, non esistono le preoccupazioni di ordine politico e sociale che hanno suggerito la scelta della perequazione integrale, ancorché ai valori standard. Rispetto a queste ultime è quindi attuata una perequazione nei limiti della sola capacità fiscale, tale da assicurare che le dotazioni di risorse non varino in modo eccessivo da territorio a territorio e, quindi, sia compatibile con una maggiore differenziazione territoriale nella composizione della spesa pubblica locale. perequazione opera, invece, con modalità sostanzialmente orizzontali, tramite trasferimenti infraregionali. Si tratta comunque di un modello congruente con lo spirito dell'articolo 119 della Costituzione. In definitiva, la ricomposizione degli strumenti sul versante sia delle entrate che delle spese si pone l'obiettivo di ottenere, allo stesso tempo, il risultato di un'ordinata responsabilizzazione finanziaria delle Regioni e degli enti locali, coniugandola con la possibilità di sviluppare, a livello regionale e locale, politiche economiche anche attraverso il ricorso alla leva fiscale. Tra gli altri principi, va messo in evidenza, in particolare, quello della territorialità, ritraibile dall'articolo 119 della Costituzione, ai fini dell'attribuzione dei gettiti, in modo da responsabilizzarne - salvo l'effetto della perequazione - le politiche territoriali nel favorire dinamiche di sviluppo autonomo. A tale proposito, in relazione in particolare all'IVA, è stato chiarito che per i servizi il luogo di consumo può essere identificato nel domicilio del soggetto fruitore finale. Questo è importante per la metodologia di locazioni delle basi imponibili e del relativo gettito sul territorio. nell'ottica dell'evoluzione temporale del sistema, è stato altresì approfondito il profilo intrinsecamente evolutivo del modello. La quota di fondo perequativo spettante a ciascuna Regione è, infatti, commisurata alla differenza tra due grandezze, una sola delle quali (il gettito dei tributi propri) è però suscettibile, in varia misura, di adeguarsi di adeguarsi automaticamente all'incremento del PIL e del livello dei prezzi, mentre l'altra (il costo standardizzato delle funzioni) non presenta analoga caratteristica intrinseca, in quanto affidata ad altri strumenti. A fronte di questo possibile esito, pertanto, il disegno di legge prescrive una periodica verifica di congruità della copertura del fabbisogno relativo alle funzioni in questione. Inoltre, l'articolo 20 prevede che i criteri di computo delle quote del fondo perequativo si applichino a regime solo dopo l'esaurirsi di una fase di transizione diretta a garantire il passaggio graduale dai valori dei trasferimenti rilevati nelle singole Regioni come media nel triennio 2006-2008, al netto delle risorse erogate in via straordinaria, ai valori determinati con i criteri dello stesso articolo 7 e che l'utilizzo dei criteri definiti dall'articolo 7 debba avvenire a partire dall'effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali degli enti locali, mediante un processo di convergenza dalla spesa storica al fabbisogno standard in un periodo di tempo sostenibile. L'altro grande capitolo del federalismo fiscale riguarda l'assetto della finanza delle Province e dei Comuni ed i relativi strumenti di entrata e spesa, e, in particolare, il ruolo di coordinamento svolto dallo Stato e dalle Regioni. A tal proposito, A tal proposito, il Capo III si sofferma sia sulla finanza degli enti locali che sulle nuove modalità di finanziamento delle città metropolitane. La scelta operata è quella di configurare un assetto della finanza locale in cui viene attribuito un ruolo significativo anche alle Regioni nel delineare schemi concreti di coordinamento della finanza degli enti locali, nel rispetto - per quanto riguarda la perequazione - dei criteri generali e delle garanzie comunque fissate nel disegno di legge di delega. In tal modo, si è chiaramente inteso individuare un punto di equilibrio tra Stato, Regioni ed enti locali, in sede di attuazione della perequazione statale all'interno di ogni territorio regionale secondo il metodo dell'intesa con gli enti locali: potranno, quindi, ridefinire la spesa e le entrate standardizzate degli enti locali secondo i criteri di riparto fissati dal legislatore statale riferiti al proprio territorio. In tema di finanziamento degli enti locali l'esame in Commissioni riunite ha apportato due modifiche rilevantissime: la prima è l'indicazione di un riferimento preciso per l'autonomia tributaria degli enti locali, ovvero gli immobili per i Comuni e il trasporto su gomma per le Province in secondo luogo, va sottolineata la previsione, alla lettera *g)* dell'articolo 11, della valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali per l'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni con particolare riferimento alla specificità dei piccoli Comuni, anche con riguardo alle loro forme associative, e dei territori montani. Non vi è chi non veda, infatti, come una applicazione del nuovo modello che non tenga conto della notevole diversificazione dimensionale e strutturale dei Comuni italiani renderebbe inapplicabile la riforma nel suo complesso. Riguardo agli interventi speciali, e quindi con riferimento all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, quinto comma, l'articolo 16 prevede che al finanziamento degli interventi in parola si provveda tramite contributi speciali dal bilancio dello Stato, finanziamento dell'Unione europea (UE) e cofinanziamenti nazionali, in base ad alcuni principi e criteri direttivi. A tale proposito si segnala l'introduzione del metodo della programmazione pluriennale per gli interventi speciali per la coesione e il Mezzogiorno, sottraendoli alla logica delle manovre finanziarie annuali. In proposito, va sottolineata la esplicita disciplina degli strumenti della fiscalità di sviluppo, anche alla luce dei più recenti orientamenti estensivi espressi dalla Corte di giustizia delle Comunità europee. In ordine alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome, l'articolo 24 prevede una forma di coordinamento realizzato chiamando tali soggetti istituzionali a concorrere tanto agli «obblighi posti dall'ordinamento comunitario» quanto agli «obiettivi di perequazione

La realizzazione di tali obblighi ed obiettivi viene demandata alle norme di attuazione degli Statuti speciali. È chiaro che nel concreto articolarsi futuro delle relazioni tra lo Stato e le Regioni a Statuto speciale si determinerà il contributo che queste saranno chiamate a fornire al disegno di perequazione, dal momento che non sono per esse stabilite regole o principi precisi, neanche per il periodo di transizione nel passaggio al nuovo regime. Venendo alla parte finale del provvedimento, una separata considerazione merita infine il problema della attuazione di una riforma di tale portata innovativa mediante una legge delega, cui dovranno seguire i relativi decreti legislativi di attuazione. Le questioni sollevate del disegno di legge in esame mostrano, infatti, che l'attuazione del federalismo fiscale presenta aspetti di notevole complessità metodologica, prima ancora che applicativa. Parecchi sono i nodi attuativi che andranno affrontati, non semplici da sciogliere, nella definizione dei canoni che regoleranno i rapporti tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali in materia di potestà tributaria, come in materia di perequazione e di coordinamento della finanza pubblica. Per il momento, il compito della delega è solo quello di stabilire, con la massima precisione possibile, i principi e criteri direttivi di carattere generale, fornendo la sola cornice dei parametri entro cui dovrà svolgersi la concreta definizione delle grandezze entro cui dovrà svolgersi la concreta definizione delle grandezze in gioco. Tra l'altro, va notato che il fatto che si tratti di una delega nel senso più aderente allo spirito della Costituzione, l'assenza di una base di ipotesi quantitative interessanti e significative hanno fatto sì che non si sia avuta fin dall'inizio una esplicitazione numerica dell'effetto delle tante variabili in gioco. Questo naturalmente sarà uno dei compiti della legislazione delegata. Saranno naturalmente i singoli decreti legislativi ad individuare, settore per settore, le conseguenze finanziare dell'attuazione della delega, una volta che saranno stati individuati i parametri e le aliquote oggetto delle scelte del Governo. La questione è talmente rilevante che proprio, e non casualmente con il contributo determinante dell'opposizione, si è prevista l'istituzione di una Commissione bicamerale *ad hoc* per l'espressione dei pareri sui vari decreti attuativi. Sul piano procedurale, è stata esplicitamente disciplinata la procedura di esame da parte del Parlamento degli schemi di decreti legislativi, e ciò al fine di garantire la massima efficacia di tale fase, di tale fase, ricorrendo alle procedure già più volte previste in sede di delega, prevedendosi, come si è detto, sia una apposita Commissione bicamerale che la salvaguardia del ruolo delle Commissioni bilancio. prevedendosi, come si è detto, sia una apposita Commissione bicamerale che la salvaguardia del ruolo delle Commissioni bilancio. Un altro punto risolto riguarda la trasparenza contabile dell'impianto proposto. Sul punto, si è partiti dalla consapevolezza della necessità di consolidamento dei conti di tutte le gestioni pubbliche interessate che, direttamente o indirettamente, fanno capo alle finanze pubbliche, consentendo il monitoraggio territoriale dei conti pubblici per macroaree (Regioni), così da costruire i valori degli aggregati finanziari di ogni singolo ente in modo coerente con l'impianto complessivo prefigurato. Diversamente, il rischio che si sarebbe corso sarebbe stato quello di non riuscire nel monitoraggio costante delle grandezze economiche di ogni Regione o ente locale creando ostacoli alla corretta determinazione della reale capacità fiscale dei singoli soggetti, con i relativi effetti sulla fissazione dei fabbisogni finanziari ed i relativi gradi di perequazione. Questo tema consente anche di operare una riflessione più ampia sulla coerenza tra il nuovo impianto dei rapporti finanziari tra i diversi livelli di governo e l'attuale configurazione normativa della decisione annuale di bilancio. Si ricorderà che più volte, nell'ambito delle ricorrenti discussioni in ordine alle ipotesi di riforma dello «strumentario» di politica finanziaria, è stata avanzata la proposta di trasformare la legge finanziaria in una legge annuale di stabilità, al fine di rendere tale strumento più coerente con la necessità di rendere la decisione annuale di bilancio più stringente rispetto all'obiettivo del rispetto dei parametri finanziari comunitari, obiettivo peraltro riaffermato dal testo in parola. Si tratta di un punto che meriterà di essere approfondito, magari in un distinto disegno di legge, al fine di rendere coerente la configurazione normativa del federalismo fiscale con la organizzazione della decisione annuale di bilancio dello Stato. Ciò consente poi L'obiettivo affermato della riduzione della pressione fiscale dei diversi livelli di governo è stato accompagnato altri versi ancora superiore. L'obiettivo affermato della riduzione della pressione fiscale dei diversi livelli di governo è stato accompagnato dalla previsione della determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale, nonché del suo riparto tra i diversi livelli di governo, anche al fine di dare garanzia ai contribuenti, gli unici veri destinatari della riforma all'esame. Anche in questo caso di tratta di una norma che anche l'opposizione ha giudicato, seppure solo in sede di prima applicazione, come indispensabile, anche se più complessa è ovviamente la sua configurazione a regime.

voglio innanzitutto dare atto al ministro Roberto Calderoli per il Governo e al relatore Antonio Azzollini per la maggioranza di avere condotto la discussione sul disegno di legge delega relativo al federalismo fiscale all'insegna di un'apertura autentica al confronto con le proposte avanzate dall'opposizione. Il Partito Democratico ha ispirato le sue proposte al disegno di legge presentato in materia, al quale si accompagna anche il disegno di legge sulla Carta delle autonomie locali. Anche gli altri Gruppi dell'opposizione hanno fornito i loro autonomi e importanti contributi. Il testo proposto all'Aula è, dunque, il risultato del lavoro delle Commissioni. È un testo diverso rispetto a quello originariamente presentato dal Governo e, nonostante il poco tempo a disposizione, il lavoro si è svolto con grande serietà, tenendo conto anche del contributo venuto dalle audizioni. Quello che viene qui presentato non è affatto un testo confuso o contraddittorio, poiché le diverse tesi si sono confrontate e sono state compiute scelte nette, in qualche caso accogliendo le proposte delle opposizioni, in qualche altro caso non accogliendole. Il nostro Gruppo nelle Commissioni riunite si è astenuto sul mandato al relatore, pur riconoscendosi in molte parti del testo attuale. Vi sono ancora punti importanti che non ci convincono e che riproporremo nella discussione in Aula. Comunque, si è aperta una strada che ci auguriamo possa concludersi, al termine del percorso parlamentare, con un testo ancora migliore, che possiamo pienamente condividere. Il metodo seguito finora nell'esame di questo disegno di legge costituisce, in questo primo scorcio di legislatura, una rara eccezione che merita di essere positivamente sottolineata, soprattutto rispetto ad un Governo che sistematicamente umilia il Parlamento, legiferando in maniera affrettata attraverso decreti-legge e questioni di fiducia e un Presidente del Consiglio che non perde occasione per negare ogni ruolo all'opposizione. Ci auguriamo che questo sia il metodo che verrà seguito anche sulle altre grandi riforme, abbandonando la contrapposizione sistematica e la campagna elettorale permanente, che non risolvono alcun problema. Il Partito Democratico è fortemente interessato all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Voglio ricordare che il centrosinistra approvò nel 2001 la riforma del Titolo V con i soli suoi voti. Successivamente il centrodestra nella legislatura che iniziò nel 2001 approvò uno stravolgimento complessivo del testo costituzionale, che venne successivamente bocciato nel referendum del 2006. Ma di questa modifica non faceva parte l'articolo 119 poiché evidentemente lo stesso schieramento che non aveva votato la riforma del 2001 lo riteneva meritevole di essere mantenuto. Da quel momento, e in particolare nella scorsa legislatura, è iniziata una fase di confronto nella quale, mano a mano, è venuta prevalendo l'idea di dare attuazione al testo costituzionale. Noi di questo siamo pienamente convinti perché è una necessità per il Paese. Si può certamente pensare di migliorare il testo del Titolo V. Noi, ad esempio, lo proponiamo, prevedendo di spostare tra le materie di legislazione esclusiva dello Stato i trasporti e la distribuzione dell'energia e introducendo un doveroso meccanismo di supremazia per il livello centrale trasversale alle materie, previo consenso del Senato federale. Ma in questo momento prevale l'esigenza di una attuazione delle norme costituzionali, come la stessa Corte costituzionale ha richiesto a più riprese, in modo particolare per l'articolo 119, anche per definire con chiarezza i rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali. il governo Prodi nella scorsa legislatura, oltre alla Carta delle autonomie locali, presentò anche il disegno di legge di attuazione dell'articolo 119 ed è stato il primo Governo a farlo dopo l'approvazione della riforma costituzionale. Dovete riconoscere, signori della maggioranza e signori del Governo, che l'alleanza tra Popolo della libertà e Lega Nord aveva presentato in campagna elettorale il cosiddetto modello lombardo, espressione dello slogan secondo cui i soldi delle tasse devono rimanere dove sono stati prelevati, a discapito di elementari principi di progressività delle imposte e di solidarietà nazionale. Ma quando il ministro Calderoli ha iniziato il percorso per giungere all'approvazione della legge, ha dovuto prendere atto che quella proposta non sarebbe mai passata, che era sbagliata e con realismo l'ha dovuta abbandonare, adottando un impianto simile a quello proposto dal centrosinistra nella scorsa legislatura. È venuto poi, pur con condizioni, il parere favorevole della Conferenza unificata e siamo arrivati a quel lavoro in Commissione di cui ho già dato atto.

ci sia uno strettissimo rapporto, anzi vorrei dire un rapporto di bruciante attualità, tra il tema che stiamo qui affrontando e la questione dell'emergenza sociale ed economica

non si fa per sventolare un vessillo di egoismo territoriale mettendo una parte del Paese contro un'altra, i Paesi che sono cresciuti di più, anche in termini di competitività, in questi anni sono quelli che hanno puntato di più sulla coesione nazionale. È quindi necessario porsi il problema di ricostruire il patto di unità nazionale, oggi fortemente messo in discussione e lacerato da divisioni profonde tra le diverse parti del Paese, a partire da un impianto nuovo di rapporti anche fiscali e finanziari tra il centro e le autonomie territoriali, e l'articolo 119 della Costituzione ce lo consente. Il federalismo fiscale non si fa per aumentare o diminuire la spesa pubblica e conseguentemente la pressione fiscale, a meno che non si segua un vecchio e deplorevole andazzo italiano

E neanche si può pensare di usare il federalismo fiscale in modo surrettizio per ridurre le protezioni sociali, per ridurre la possibilità da parte di Regioni ed enti locali di far fronte con i propri mezzi alla necessità di finanziare le prestazioni, mentre è giusto lasciare, naturalmente, a quegli enti la possibilità di migliorare le prestazioni agendo sulle loro leve di autonomia fiscale. Il federalismo fiscale non si fa neanche per decentrare funzioni amministrative dal centro verso le Regioni e le autonomie locali, perché quella è la funzione della Carta delle autonomie locali e in modo particolare dell'articolo 118 della Costituzione, che prevede una riattribuzione delle funzioni pubbliche in base al principio di sussidiarietà: tutte quelle che sono possibili al livello più vicino ai cittadini, mantenendo al centro solo quelle che non si possono diversamente allocare. Il rapporto con la crisi è molto forte e molto stringente particolarmente Il primo riguarda la necessità per il nostro Paese, come hanno fatto e stanno facendo pressoché tutti gli altri Paesi più economicamente sviluppati, di fare politiche espansive di bilancio, perché il rigore nei conti pubblici, a cui noi crediamo e che ha ispirato anche le politiche del nostro precedente Governo, lo si persegue sostenendo soprattutto la crescita economica

vuol dire parlare della possibilità - certo non oggi, ma nel momento in cui questo provvedimento darà i suoi frutti - di cambiare lo Stato italiano, di cambiare la pubblica amministrazione, rendendola più vicina ai cittadini significa rendere più autonomi i livelli territoriali locali e regionali rispetto alle scelte che devono compiere sia in materia di entrate, sia in materia di spese. Ricordiamo che questa tendenza al decentramento delle funzioni e anche dell'autonomia tributaria non è propria solo degli Stati classicamente federali (Stati Uniti, Canada, Germania, Svizzera, Australia), ma negli ultimi anni è diventata propria anche di grandi Stati unitari che pure si stanno articolando fortemente al loro interno, come il Regno Unito, la Spagna, il Belgio. La stessa Francia, che pure ha una tradizione fortemente centralistica, ha negli anni scorsi promosso forti riforme proprio in materia di sostegno alle autonomie locali

noi siamo pienamente convinti che un'azione di decentramento e di rafforzamento delle autonomie serve a rendere più efficiente lo Stato e quindi a dare un'arma in più alla possibilità di combattere la crisi in atto. Da queste Da queste considerazioni di carattere generale consentitemi di venire subito ai tre problemi fondamentali, preliminari rispetto al testo, che i colleghi che hanno partecipato al dibattito conoscono bene, perché li abbiamo posti più volte e che a noi paiono ancora irrisolti nel momento in cui arriviamo in quest'Aula. Dico subito che ci auguriamo che su ciascuno di questi problemi già dal dibattito in Aula possano venire da parte del Governo e della maggioranza chiarimenti per noi indispensabili

Signori della maggioranza e del Governo, vi pare possibile che di fronte alle nostre reiterate richieste di avere le simulazioni circa gli effetti prevedibili dal punto di vista finanziario di questo disegno di legge o quantomeno un intervento chiarificatore del Governo sull'impatto di questa legge sull'attuale situazione di grave crisi economica, non abbiamo avuto altro che un silenzio? Un silenzio che riteniamo grave e inaccettabile. Certo, c'è una responsabilità collegiale del Governo ma c'è soprattutto un Ministro dell'economia, che tra l'altro è primo firmatario del disegno di legge in questione, che è il vero convitato di pietra di questa discussione, che sta assumendo un atteggiamento di silenzio assordante su questi temi. Noi ci auguriamo che nel corso della discussione generale in quest'Aula e nella replica del Governo anche il ministro Tremonti voglia degnarsi di venire qui e prendere la parola.

la parte della Costituzione relativa al trasferimento dei poteri verso i livelli più vicini ai cittadini, non basta l'attuazione dell'articolo 119, che pure è importante. Occorre attuare anche gli altri articoli collegati: in particolare, il 114, il 117 e il 118, che ho già illustrato prima, per evitare che nel migliore dei casi diamo nuovo carburante ad una macchina vecchia, ad un motore vecchio, quale è l'attuale organizzazione dei poteri pubblici italiana, che va cambiata nel profondo anche per sostenere la crescita del Paese. Dobbiamo allora accompagnare al federalismo fiscale la Carta delle autonomie locali. A tal proposito, il ministro Maroni non ci ha convinto quando in Commissione ha riferito che tra qualche settimana il Governo approverà il testo. Qualche settimana può voler dire anche molti mesi; vogliamo sapere quando questo

per il mancato gettito dell'ICI sull'abitazione principale non gli è stato ancora trasferito. Il Senato ha approvato un ordine del giorno su questo tema. Noi chiediamo che il Governo, così come sul punto precedente inerente gli investimenti degli enti locali, assuma in questa sede precisi impegni affinché quell'ordine del giorno venga Vengo ora all'illustrazione molto rapida dei sette punti sui quali le nostre proposte sono state raccolte dal testo attuale e dei cinque punti su cui le nostre

per l'attuazione del federalismo fiscale, una proposta contenuta nel nostro disegno di legge. Noi insisteremo perché il comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali

la Segreteria tecnica, venga almeno in parte nominato dalla Commissione parlamentare, attraverso figure di tecnici autorevoli e indipendenti, affinché questo organismo diventi una vera e propria Il secondo punto riguarda il patto di convergenza, la proposta fondamentale del nostro disegno di legge. Insieme al passaggio dalla spesa storica ai costi standard, vi deve essere anche l'impegno a non fotografare l'attuale situazione di assurda disparità nell'offerta di servizi tra le varie parti del Paese, ad esempio

del patto di convergenza, dell'indicazione dei saldi da rispettare, nonché di un obiettivo di pressione fiscale programmato che tenga conto dell'autonomia tributaria dei vari livelli di governo. Occorre fare attenzione perché Banca d'Italia, ISTAT e Corte dei conti ci hanno messo in guardia rispetto al fatto che questo processo non deve aumentare la pressione fiscale. Noi siamo d'accordo, come ha già detto il relatore

riguarda l'accoglimento del termine di 12 mesi per l'adozione del primo decreto legislativo, avviando così un processo che altrimenti non aveva termine. Faccio presente che un'altra delle modifiche è stata l'avere stabilito che la fase transitoria durerà comunque cinque anni e non «un tempo sostenibile», come prima era scritto. Vengo invece ai punti su cui abbiamo avuto risposta parziale e che consideriamo ancora aperti, alcuni di questi totalmente aperti e sui quali faremo battaglia parlamentare per avere le risposte dovute e anche per migliorare ulteriormente il testo. riguarda l'introduzione del principio del finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite alle autonomie territoriali. Si tratta di un principio importantissimo, ma bisogna stare attenti che a questo principio corrisponda anche il funzionamento dei fondi perequativi. definizione dell'ambito di autonomia tributaria delle Regioni. È molto importante avere chiarito nel testo che il principio di territorialità delle imposte, come prevede la Costituzione, si riferisce solo ai tributi regionali e locali e alla compartecipazione erariale, e non ai grandi tributi erariali. Questa è una questione fondamentale: se fosse passata l'idea di una appropriazione territoriale del gettito dei tributi erariali, non avremmo più i presupposti di uno Stato unitario. Crediamo quindi, avendo contribuito a chiarire questo punto, di aver reso un servizio a tutta la nostra istituzione, il Parlamento italiano, perché in tal modo chiariamo bene che vogliamo

funzioni di comuni e Province, ancorché nella fase transitoria, e Roma Capitale. Come sanno il Ministro e la maggioranza, abbiamo chiesto di stralciare queste parti e di collocarle nella Carta delle autonomie locali. è comunque necessario riscrivere la parte sulle funzioni, in modo tale che sia chiaro che un'eventuale delimitazione eccessiva di tali funzioni non pregiudica la discussione in sede di Carta delle autonomie locali sulle funzioni fondamentali, e inserire nella legge anche il tema delle Città metropolitane, perché lo riteniamo assolutamente necessario. Con questo ho concluso l'illustrazione del testo proposto all'Assemblea dalle Commissioni. Qualcuno, maliziosamente, ha voluto insinuare che il nostro atteggiamento costruttivo sarebbe dovuto alla volontà di insinuarci nella maggioranza per creare contraddizione tra le sue diverse componenti. Qualcun altro, meno benevolmente, ci ha attribuito l'intento di strizzare l'occhio alla Lega Nord per ragioni strumentali. Siamo alternativi alla Lega Nord e alle altre forze che compongono la maggioranza e lo dimostrano le tante battaglie parlamentari, anche molto accese, che conduciamo su molte proposte del Governo, alcune delle quali espressamente volute dalla Lega Nord. Questo però non ci impedisce, su grandi questioni istituzionali come questa, di avanzare proposte con l'intento di dar vita a provvedimenti condivisi. Il nostro atteggiamento conclusivo in questa Aula dipenderà solo dall'accoglimento o meno di proposte che consideriamo importanti, oltre alle tante già contenute nel testo, perché il nostro intento è uno solo, e lo dico agli osservatori maliziosi e interessati: contribuire a dare al Paese una buona legge sul federalismo fiscale, poiché pensiamo che di una buona legge in questa importante materia il Paese abbia davvero bisogno.

e non per ragioni di forma, dare atto sia del lavoro svolto dal ministro Calderoli, sia politicamente dare atto alla Lega di avere introdotto un tema ed un dibattito sul piano politico di rilevanza strategica per il futuro del Paese. Lo voglio dire senza alcuna riserva mentale, perché riteniamo che l'approccio corretto su questo tema sotto il profilo metodologico sia il confronto parlamentare, avvenuto in Commissione e che avviene in Aula, al di là delle questioni di merito che nella sede propria, cioè la discussione generale sul provvedimento, avremo modo di illustrare, ci riserviamo di dare una valutazione definitiva rispetto al voto di astensione che abbiamo dichiarato in Commissione.

le norme costituzionali rendendo effettive le previsioni che oggi lo sono solo in virtù della sistematica interpretazione della Corte costituzionale in ordine ai rapporti tra Stato, Regioni ed autonomie e, quindi, avendo scelto un percorso minimalista, cioè di attuazione di una delle norme che regolano il rapporto così come

un disegno di legge ordinario che, peraltro, contiene una serie di deleghe al Governo; quindi è chiaro che questo è il binario che ci è stato dato per il confronto e a questo dobbiamo attenerci. Per tale ragione ci permettiamo di fare una serie di rilievi che riteniamo fondati e che sottoponiamo all'esame dei colleghi con assoluta serenità, partendo dal presupposto che il nostro interesse è che da questo confronto parlamentare esca un provvedimento che sia in linea con i principi e con le norme contenute nell'articolo 119 della Costituzione. Per questa ragione, signor Presidente, riteniamo che vi siano alcuni profili di contrasto con l'articolo 76 della Costituzione. Il primo, dal nostro punto di vista, riguarda le modalità di finanziamento delle funzioni amministrative attribuite a Regioni ed enti locali nella parte in cui si fa riferimento a tipologie distinte di funzioni senza che le stesse siano individuate. la delega sul federalismo fiscale non disciplina solo il contenuto dell'articolo 119, ma, dovendo necessariamente individuare i livelli delle prestazioni essenziali e quelle previste dall'articolo 117, comma 2, dovrebbe contenere almeno l'indicazione, la tipologia e le caratteristiche proprie per consentire poi al Governo di quantificare con esattezza - perché questo impone l'articolo 81 della Costituzione - le risorse necessarie per la copertura.

lo Stato desse copertura integrale con proprie risorse a carico della fiscalità generale, proprio per distinguere in maniera netta chi fa o che cosa fa: cosa deve fare lo Stato, cosa devono fare le Regioni e cosa deve fare il sistema delle autonomie. A ciò vorrei anche aggiungere che

con lo spirito e la norma dell'articolo 76 della Costituzione; e ciò sotto due profili: quello della genericità dell'oggetto e quello della irragionevolezza del termine per l'esercizio della delega, che è prolungato in modo da sovrapporsi ad un'intera legislatura. Inoltre, trattandosi di deleghe correttive, si parte dal presupposto che il tipo di correzione intervenga solo su aspetti marginali e non profondi e sostanziali del testo, il la dice lunga sul livello di genericità della delega stessa e sull'impossibilità, seguendo il metodo che la maggioranza ha voluto adottare, di poter disporre di dati e norme di riferimento certe e di un assetto istituzionale che sia, così come prevede l'articolo 119 della Costituzione, integralmente finanziato con le risorse ivi disciplinate. Ci sembra peraltro una forzatura sotto il profilo costituzionale l'idea che la commissione disciplinata dall'articolo 5 della delega, la cosiddetta commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, possa sostanzialmente sostituirsi al Parlamento nella determinazione delle risorse e delle modalità attraverso cui si finanzia il fondo perequativo e le altre attività connesse all'attuazione del federalismo fiscale. L'articolo 119 della Costituzione recita che il fondo perequativo è istituito con legge dello Stato, il che sta a significare che esiste un'unica sovranità parlamentare per la definizione delle quantità e della qualità degli interventi che si attuano attraverso il fondo perequativo. Peraltro, com'è noto, la materia della perequazione è di competenza esclusiva dello Stato;

particolare al Parlamento, che può delegare una parte della sua sovranità solo ed esclusivamente al Governo, cioè può ad esso delegare l'esercizio del potere normativo in via eccezionale secondo le regole dell'articolo 76 della Costituzione, non ad altri organi come il comitato permanente. norma risiede nel fatto che è lo strumento che fa la differenza nell'ambito della ricostruzione di un equilibrio sociale, rispetto alle ampie forme di decentramento fiscale che si introducono con tale provvedimento:

A questo voglio aggiungere che, proprio perché c'è una riserva di legge assoluta su questo tema, la Costituzione prevede, come unico criterio per la gestione e l'erogazione delle risorse previste in questo fondo, la capacità fiscale per abitante, proprio a sottolineare la circostanza che il legislatore statale non ha neanche un potere discrezionale nella valutazione delle modalità con cui destinare

Credo che dovremmo anche fare una riflessione per quanto riguarda alcuni aspetti del fondo perequativo con riferimento alla circostanza che gli articoli 9 e 13 della legge delega sul federalismo fiscale prevedono che la destinazione delle risorse del fondo perequativo al sistema delle autonomie locali, cioè ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane, eccetera,

secondo luogo, il fondo perequativo infrastrutturale è in netta violazione delle prerogative previste dagli Statuti. Mi riferisco in modo particolare all'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana 25 del testo del disegno di legge, alla riserva prevista espressamente dall'articolo 43 dello Statuto siciliano (ma credo che sia norma comune a tutti gli Statuti speciali), in virtù della quale le disposizioni che regolano i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni a Statuto speciale sono norme pattizie che passano attraverso le norme di attuazione e la Commissione paritetica. principio, si viola un caposaldo del federalismo che è stato anticipato dalle Regioni a Statuto speciale. Per queste ragioni, noi riteniamo opportuno approvare la questione pregiudiziale per motivi

momenti del dibattito e anche del voto sul provvedimento, ma certamente non incidono sulla compatibilità del disegno di legge con le norme costituzionali.

Non mi sembra che vi siano argomenti per sostenere questo assunto e devo dire che di principi e criteri direttivi è ricca la delega. Certamente una delega può essere più o meno dettagliata, ma il dettaglio che contiene il disegno di legge è più che sufficiente per contestare l'affermazione secondo la quale si tratta di una delega in bianco. argomenti sollevati è che la legge di delega dovrebbe contenere anche riferimenti precisi alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali, invece verrebbero in qualche modo assunti al di fuori del processo di attuazione e di deliberazione sul federalismo fiscale. Certamente è così e non può essere che così, perché le norme sulle funzioni fondamentali e sui livelli essenziali sono norme di diritto sostanziale, sono sparse nel nostro ordinamento in vari provvedimenti, sono scritte nell'attuale testo unico, sono scritte nelle leggi riguardanti i vari settori nei quali si esplica la competenza concorrente o esclusiva delle Regioni o l'esercizio delle funzioni degli enti locali. Certamente esiste un'esigenza, che non riguarda il livello costituzionale, di riordinare questo complesso di norme proprio per poter meglio attuale il federalismo fiscale. Su questa linea è impegnato

all'attuazione del federalismo fiscale. Lo stesso si può dire per le deleghe correttive: è evidente che la formula utilizzata nel testo del disegno di legge è usuale e tralatizia,

la potestà correttiva venisse utilizzata per stravolgere una delega già esercitata o per compiere scelte diverse o antitetiche (come si è cercato di fare per alcune deleghe nel passaggio dal Governo Berlusconi al Governo Prodi), si tratterebbe di un esercizio improprio del potere correttivo di delega. Altra obiezione che mi sembra meritevole di contestazione è quella sul fondo perequativo: ritengo che non vi sia alcuna violazione dei principi costituzionali, ma è evidente che il fondo perequativo ordinario, così come recita l'articolo 119, viene stabilito sulla base della capacità fiscale delle singole comunità regionali ed è la stessa norma norma costituzionale ad escludere che vi siano vincoli di destinazione. Quindi, l'uso che se ne farà - e dunque la distribuzione di questo fondo per l'una o per l'altra funzione, per l'una o per l'altra competenza non può che essere demandato all'organo regionale, che è il punto di riferimento del federalismo fiscale. Infine, sulle Regioni a Statuto speciale ritengo vi sia stato un passaggio fortemente migliorativo nel testo del disegno di legge che qui oggi esaminiamo e non vi sia alcuna violazione delle prerogative di tali Regioni. delle prerogative di tali Regioni. Ricordo, infatti, che quelle già esistenti in base agli Statuti speciali vengono conservate e finanziate come nel passato; il problema si pone per quelle ulteriori competenze e prerogative che la novella del

complicato, certamente non vi è alcuna possibilità, almeno sotto il profilo di una delega correttamente esercitata, di incidere in maniera inappropriata sulle competenze delle Regioni a Statuto speciale.

che crea rilevanti problemi di attuazione e li creerà anche in futuro, ma è una legge che serve per dare finalmente attuazione ad un grande principio

discuterlo, guardarne gli aspetti innovativi e cercare ancora di migliorarlo nel corso dei lavori parlamentari. Siamo convinti che il Paese abbia bisogno di

molto intensamente alla discussione in Commissione e sono presenti anche in Aula. Si direbbe dovere istituzionale; ed è stato così per il lavoro svolto in Commissione con la più assidua presenza, in particolare del ministro Calderoli; non è così per quanto riguarda naturalmente la presenza del ministro Tremonti. Vorrei sottolinearlo questo punto. Colleghi, per cortesia, invito chi non intende rimanere in Aula a uscire per poter permettere alla collega Incostante di fare il suo intervento. Volevo sottolineare l'assenza - come già detto - del ministro Tremonti; personalmente la reputo davvero inaccettabile. Credo che i membri del Governo tutti, per la loro responsabilità collegiale, dovrebbero sentire questo peso e questa assenza. Non è una questione speciosa, ma di sostanza: il ministro Tremonti è il primo firmatario di questo provvedimento; siamo nel pieno di una crisi economica e finanziaria di notevoli proporzioni; abbiamo chiesto al Ministero dell'economia di avere dati, anche se macro e di scenario, sulla ricaduta di questo provvedimento, ma ancora una volta questo elemento rimane senza risposta. Dico ai Ministri più sensibili, che hanno lavorato di prendere nota di questa mancata risposta da parte della maggioranza. Si tratta di una mancata risposta politica, sostanzialmente anche per l'atteggiamento indifferente del ministro Tremonti rispetto alle richieste di tre Commissioni riunite e del Parlamento. Credo che ciò condizionerà anche il nostro atteggiamento nel prosieguo dei lavori. Voglio dirlo molto francamente: sicuramente ci sarebbe dovuto essere il conforto del Ministero dell'economia su questioni che ci stanno molto a cuore

Venendo al merito delle questioni, credo che la nostra proposta abbia potuto mettere in campo alcuni aspetti migliorativi del disegno di legge in esame e sicuramente ritengo che il lavoro fatto sia stato importante, in quanto ha dimostrato come qualche volta, se all'arroganza di chi governa si sostituisce la capacità di dialogo, forse il Parlamento viene messo in condizioni di fare davvero un lavoro positivo.

nel merito. Questa è la considerazione cui tengo di più: noi dobbiamo evitare che i decreti attuativi, sui quali abbiamo un forte sentore che invece il ministro Tremonti sarà molto attivo, diventino dopo questa legge delega uno strumento per diminuire ancora di più l'eguaglianza tra i territori, per aumentare i divari per diminuire anche la capacità e la qualità dei servizi dei territori a bassa capacità fiscale perché non è detto e scontato che, rispetto alle risorse inefficienti, necessariamente la spesa pubblica si possa riconvertire in qualità; non è detto che la scelta non possa essere quella, invece, di diminuire la qualità dei servizi e perfino il loro numero, arrivando a uno stato minimo. minimo. Il rischio è che invece di fare del federalismo fiscale, come noi abbiamo creduto e continuiamo a credere, uno strumento di efficienza, di sviluppo e di qualità della spesa pubblica, possa diventare uno strumento di rottura tra i territori che vengono così lasciati al loro destino, soprattutto nell'ambito di una crisi economica. Vorrei ripetere le affermazioni del presidente Vitaletti, che ha presieduto l'Alta commissione

un momento in cui gli effetti sconvolgenti della globalizzazione» - e oggi si potrebbe dire all'interno di questa crisi economica e finanziaria - «e il richiamo alla necessità della riduzione della sovranità fiscale nazionale spingono al coordinamento delle misure sovranazionali» - come accade negli ultimi tempi - «è arduo trovare una modalità di attuazione del federalismo fiscale, che si scontra sicuramente con margini di decentramento interno ristretti

tanto hanno contribuito ad ascoltare le nostre posizioni e a migliorarle rispetto ai temi del Mezzogiorno. Insisto al riguardo perché bisogna fare in modo, anche in queste ultime ore di lavoro, che tali questioni siano al centro della nostra attenzione.

«Ci sono stati uomini illuminati del Nord che hanno lavorato per il Mezzogiorno. Non è il caso quindi di rimettere in campo vecchie e deleterie contrapposizioni tra Nord e Sud, né presentare nuove sordità verso le esigenze meridionali», così come ha fatto questo Governo invece sui fondi FAS. «Noi dobbiamo interpretare un sentimento di unità nazionale vivo nel Paese, un patrimonio che va coltivato nella consapevolezza inderogabile dei valori della Costituzione». Il Mezzogiorno dovrà essere all'altezza di questa sfida, migliorare il suo tessuto democratico, superare le sue inefficienze, progettare e dare soluzione ai problemi del vivere civile - e per questo sono d'accordo sulle misure previste

e contro la criminalità organizzata e puntare a politiche strutturali per il Mezzogiorno. Solo in questo quadro sarà credibile il decentramento fiscale e l'attuazione di una riforma costituzionale da noi fortemente voluta nel segno della cooperazione, del decentramento e della responsabilità, ma non della rottura della nostra unità nazionale.

Quindi, il problema non è questo. Il problema è piuttosto che il Governo deve lavorare, prendere decisioni, andare avanti e non perdere tempo. Del resto, noi qui siamo talmente pochi che non credo si possa bacchettare un Ministro che sta lavorando per il solo fatto che in questo momento non ascolta i nostri sussulti.

La legge delega è stata accusata di non quantificare i costi del federalismo. Potremmo rispondere che non si possono nemmeno, al momento, quantificare le entrate nuove che produrrà o i minori balzelli che potrebbero gravare sulle spalle dei cittadini. Certo, si può già dire che la norma è nata e si svilupperà nei decreti legislativi da emanare insieme a coloro che ne sono i principali destinatari. Credo che il loro consenso di massima sia già la garanzia di una cosa fatta bene, a vantaggio di tutti, che porterà il nostro Paese ad avere una migliore amministrazione della cosa pubblica. Un obiettivo non da poco per ricostituire il legame di fiducia con i cittadini; un legame che in certi momenti è mancato e che si concretizzerà proprio nei luoghi - Regioni, aree metropolitane, Comuni - dove lo Stato è più vicino alla gente.

discussione rappresenta un atto dovuto nel lento, ma ineludibile, processo di attuazione di quella parte della Costituzione che disegna la Repubblica italiana come Stato regionale. Già in passato vi furono tentativi non sempre nobili che indussero a ritardare la realizzazione dei Parlamenti regionali. Certamente vi influirono le differenti situazioni economiche e strutturali che caratterizzano l'Italia, ma anche

Ripercorrendo la storia, osserviamo che per molti anni si sono avuti ingenti trasferimenti di risorse nel tentativo di compensare gli svantaggi tra le varie realtà territoriali. Gli strumenti e le modalità con cui questo obiettivo è stato ricercato hanno però notevolmente ridotto l'efficacia di tali investimenti e il beneficio per i destinatari. i destinatari. Ora è necessario modificare l'impostazione di fondo della gestione delle risorse che lo Stato ripartisce, con un duplice obiettivo: restituire ad ogni comunità locale la propria potenzialità di crescita e rendere efficace l'intervento perequativo, di modo che tutta l'Italia possa godere di standard elevati ed omogenei di servizi pubblici e di infrastrutture. che richiede oggi il popolo italiano, tutto, che si è espresso con chiarezza sul federalismo con il *referendum* approvato nel 2001, che modificava il Titolo V della Costituzione. Le modifiche introdotte rispetto al vecchio testo costituzionale sono numerose e riguardano, tra l'altro, la ripartizione dei poteri legislativi e di amministrazione tra i diversi livelli di governo presenti in Italia, i mezzi di finanziamento di Regioni ed enti locali; le regole di perequazione e la possibilità di forme di autonomia differenziata per le Regioni a statuto ordinario. La Costituzione ha una sua valenza aggiuntiva; essa concorre, infatti, a fissare quei giudizi di valore che consentono di costruire il ponte tra la possibile neutralità della teoria e le scelte concrete dell'azione politica. Oggi, il momento economico e sociale che attraversiamo rende inevitabile il federalismo anche sul piano fiscale; non possiamo ripetere gli errori del passato, non abbiamo più le risorse di un tempo, anche se forse quel Titolo V della Costituzione, ministro Calderoli, va pietosamente rivisto, perché non è così efficiente, né soprattutto efficace ed ingenera molta confusione: da ex consigliere regionale posso dire che in certi casi causava anche paralisi nelle scelte,

sarà chiamato a realizzare questa delicata riforma e a dare a Regioni, Comuni e Città metropolitane gli strumenti di autonomia a cui hanno diritto, si avverte pervasivo il principio di sussidiarietà, mentre la solidarietà nazionale viene assicurata da quei principi insiti nella Costituzione e spiega la propria forza unificante. Il disegno di legge delega che il Governo ha varato nasce con la precisa volontà di essere condiviso nel modo più ampio possibile. Esso ha già avuto in sede di stesura il consenso di massima da parte della Conferenza unificata, ma non basta: il comma 4 dell'articolo 2 del testo in esame dispone che il Governo assicuri, nella predisposizione dei decreti legislativi che entro due anni dovranno dare le ali al progetto federalista, piena collaborazione con le Regioni e con gli enti locali, anche al fine di condividere la definizione dei livelli essenziali di assistenza, dei livelli essenziali delle prestazioni e la determinazione dei bisogni

quanto previsto dalla legge. Il testo che il Governo ci chiama ad approvare garantisce, attraverso il fondo perequativo, che i divari in termini di entrate debbano essere ridotti. Siamo di fronte, dunque, ad un modello di federalismo fiscale di tipo solidaristico e cooperativo piuttosto che marcatamente competitivo. Certo, questo significherà comunque la necessità, per chi amministra a livello regionale e locale, di superare una mentalità vecchia,

che è stato oggetto dell'intervento della collega che mi ha preceduta, ripeto che non possiamo rispondere in questo momento né su quante

il Governo ha presentato una sua proposta, c'è stato un dialogo, un confronto; il testo che è entrato in Commissione ne è uscito diverso. Noi pensiamo sia uscito un testo migliore rispetto a quello originario; dovremo

confrontati nel merito, come si deve fare in un'aula parlamentare su provvedimenti importanti come questo.

colleghi, per noi misurarci e confrontarci non è stata una cosa semplice; abbiamo presentato anche noi un disegno di legge ma eravamo partiti da

seguire la nostra strada in questo momento, come ci ha detto anche il ministro Calderoli e il presidente Azzollini, poteva significare rimandare nel tempo un intervento che invece può essere nell'interesse del Paese e che poi ha bisogno di provvedimenti attuativi. che era molto più utile stare al confronto e misurarsi fino in fondo su questo versante e abbiamo deciso di scegliere questa strada. Credo che abbiamo fatto una cosa giusta.

non riuscire a dare certezze, garanzie e risposte appropriate, puntuali e precise è un limite.

che ci siano mai state nel mondo ed il Ministro dell'economia è sicuramente impegnato con serietà nell'interesse del Paese e di tutti noi,

che si è manifestato ed accentuato recentemente. Il cittadino, cioè, vuole sempre più essere conscio, da un lato, di come vengono spesi i quattrini che paga in imposte e, dall'altro, la territorialità dell'imposta, che meriterebbe naturalmente accenni molto più approfonditi, è comunque un elemento che tanto la Costituzione, quanto, anche in questo caso, la sensibilità comune, rendono parte integrante del disegno di legge

sui costi standard*.* Anche questa è una rivoluzione copernicana, che mette in luce un approccio totalmente diverso, diametralmente opposto rispetto a quello cui fino adesso, in questo Paese, si era abituati

Altrettanto importante è l'approccio che ha il disegno di legge delega sulla questione della perequazione. Ebbene, è una perequazione verticale ed è anche previsto dalle modifiche che il Comitato ristretto delle Commissioni ha apportato.

più opportuna una perequazione orizzontale, che metta nella giusta competizione gli enti locali, però è inutile che stiamo a discutere di qualcosa che, nella realtà dei fatti, a livello costituzionale è già predeterminato: ovviamente, è all'interno dell'alveo costituzionale che dobbiamo intervenire. Comunque sia, il fatto che la perequazione sia studiata e regolata in diversi aspetti e che rimangano sotto traccia i contributi dei vari enti locali e delle Regioni al fondo perequativo

in senso negativo ma in senso esattamente positivo. Ho sentito in qualche intervento poc'anzi parlare dell'approccio che dovrebbe vedere solamente, secondo il parere di alcuni, la fiscalità statale come elemento di costituzione dei fondi perequativi: credo

il vivere ed il sentire comune dei cittadini, dovremmo definirli enti dello sperpero, dell'inefficienza o peggio ancora: credo che anche questo sia un sintomo di grande voglia di equità; un'equità che

di potere essere in grado di autonomamente svolgere le proprie funzioni. L'insieme di questo provvedimento dà spazio ed ascolto a queste voci che credo dobbiamo ascoltare perché il Paese può cambiare e migliorare solamente se intraprende questa strada. *(Applausi

Vorrei incentrare quindi il mio breve intervento sulle questioni aperte, oggetto della nostra proposta emendativa per il confronto in Aula, con una sola premessa. Stiamo per dare attuazione all'articolo 119 della Costituzione che, per convenzione ormai generalizzata, chiamiamo del federalismo fiscale anche se, detto per inciso, l'articolo si riferisce all'autonomia finanziaria di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

votata nel 2001 e confermata da una *referendum* popolare. Non sottolineo questo aspetto per rivendicare, Ministro, una sorta di primogenitura. Spetta semmai al centrodestra spiegare ai cittadini perché nel quinquennio 2001-2006 non hanno dato attuazione a questi articoli. Abbiamo già perso troppo tempo. Ma l'ho sottolineato per richiamare un filo rosso che guida in modo coerente la nostra azione politica e legislativa su tutta questa materia. È quindi, con grande serenità e con proposte convinte che abbiamo accettato il confronto con il Governo.

vorrei dire che questa dovrebbe essere la normalità del confronto democratico in una democrazia matura; speriamo che questo sia l'inizio di un ritorno alla normalità del confronto democratico.

affonda le sue radici in una lunga tradizione cui mi sento orgogliosamente di appartenere, quella dell'autonomismo solidarista e solidale,

in grado anche di mettere la parola fine al contenzioso permanente che abbiamo registrato in questi anni e sul quale la stessa Corte costituzionale si è pronunciata più volte, chiedendo proprio al legislatore ed a tutti noi di fare chiarezza. Per questo avremmo anche preferito cominciare dalla testa invece che dalla coda, cioè dal riordino del sistema delle autonomie, perché è proprio con esso che noi possiamo conseguire l'obiettivo più alto, caro Ministro, quello di rendere il nostro apparato pubblico moderno, efficiente e trasparente, che è il vero scopo della nostra azione.

un apparato complessivo di autonomie locali non riordinato, e quindi vecchio e pieno di contraddizioni, rischieremmo

dei due provvedimenti per vedere insieme il sistema delle coerenze), ma neanche del fatto che egli ci abbia prefigurato cinque provvedimenti e cioè una materia trattata in modo disorganico. Tale carenza

in un contesto che vuole essere solamente fiscale, delle norme su Roma capitale.

ministro Tremonti oggi manchi perché si trova a Bruxelles: questo va da sé. Il problema è che egli è mancato in tutti i mesi in cui abbiamo trattato questa materia delegando totalmente al ministro Calderoli.

Signora Presidente, io parlo giunto ormai al quinto giorno di sciopero della fame mentre altre 250 persone, tra le quali

il presidente Villari, l'onorevole Beltrandi e l'onorevole Sardelli. Sto parlando della Commissione di vigilanza in particolare sul servizio radiotelevisivo pubblico che, come si legge stamani sul «Corriere della Sera», è in una fase di stallo oggettivo e irrevocabile: sono parole del Presidente del Senato. Ebbene, cosa si propone però per impedire che tutto ciò vada avanti? Si propongono delle soluzioni che, se portate avanti, creeranno dei precedenti gravissimi dal punto di vista del rispetto della legalità costituzionale in questo Paese.

all'ordine dei nostri lavori, per la necessità di riportare all'attenzione delle massime cariche dello Stato il rispetto della Costituzione.

di accordare al terrorista Cesare Battisti lo *status* di rifugiato politico. Come Italia dei Valori, riteniamo che la decisione sia di una gravità estrema e che possa, se non compromettere, almeno duramente provare i rapporti ottimi che il nostro Paese ha costantemente intrattenuto con il Brasile. Sempre ieri, e poi di nuovo questa mattina, mi sono incatenato davanti all'ambasciata brasiliana, mentre una delegazione dell'Italia dei Valori ha consegnato all'ambasciatore brasiliano qui in Italia la mozione a firma dell'Italia dei Valori e sostenuta anche da altri colleghi di ogni forza politica, La mia protesta, il mio segno forte, durerà finché all'*impasse* diplomatica, nell'affronto verso le istituzioni italiane, con il tentativo di screditare il nuovo sistema giudiziario, non si troverà una soluzione ragionevole. Credo che tutti i colleghi condividano - come hanno già fatto giovedì - questa nostra iniziativa: l'unica soluzione ragionevole è l'estradizione di un terrorista, che si chiama Battisti e che oggi un Paese come il Brasile sta addirittura Osserviamo che già il Governo brasiliano sembra accogliere, benché in minima parte, le numerose proteste e le svariate richieste, pervenute anche da parte del nostro capo dello Stato, Napolitano, che accogliamo in pieno (come ha recitato, credo, l'intero arco istituzionale, a partire dal Popolo della Libertà,

rappresentato addirittura in Brasile come un rifugiato politico, rappresenta per l'intero arco istituzionale un'offesa al nostro Paese e al nostro Capo dello Stato. Continueremo a combattere contro un condannato per quattro omicidi

del Presidente del Brasile è sicuramente uno schiaffo alle nostre istituzioni. Il Presidente della Repubblica italiana era intervenuto, come è intervenuto il presidente della Camera Fini.

Il problema di fondo è questo, però voglio riferire un episodio che alcuni grandi quotidiani hanno riportato. In questi giorni alcuni terroristi rossi (dico "rossi" perché appartenenti a gruppi politici ben riconosciuti) hanno chiesto - o sembra che stiano per chiedere - all'INPS la pensione di vecchiaia. Questo è uno scandalo che non viene riportato